umane in favore del Mezzogiorno, il programma Next generation EU è il più ambizioso progetto di investimenti che l'Unione europea abbia mai messo in campo. Un'occasione unica non solo per far rialzare il nostro Paese duramente colpito dalla crisi pandemica, ma anche e soprattutto per ridare centralità all'Italia nel panorama economico internazionale. In tale contesto assume particolare rilevanza anche il rilancio del Mezzogiorno, a partire dall'utilizzo di queste risorse per colmare il divario Nord-Sud, così come richiesto dall'Europa. Ministra, apprezziamo la sua attenzione e la ringraziamo per il suo prezioso lavoro e per la disponibilità con cui ha ricevuto e ascoltato la delegazione dei sindaci del *Recovery* Sud, ma ora attendiamo misure concrete dal Governo e che sia dato al Sud ciò che gli spetta. Un Sud Un Sud da anni fortemente disallineato rispetto al Centro-Nord sul piano economico, produttivo, sociale e, come abbiamo potuto purtroppo accertare in questi ultimi mesi, anche sanitario. Un esempio tra i tanti è la mia Regione, la Calabria e, in particolare, la provincia di Cosenza, che in questi giorni vive il momento peggiore dall'esplosione della pandemia, con un significativo e crescente aumento dei contagi e dei decessi. Un'Italia a due velocità, con un Mezzogiorno sempre più distante dal resto della Nazione, non è più sostenibile per la stabilità finanziaria del Paese, né giustificabile alla luce delle ingenti risorse che saranno destinate al Sud e soprattutto per la strategica posizione geografica che essa assume nel contesto europeo e internazionale. Inoltre, è evidente che il piano delle assunzioni previste per i Comuni del Sud è nettamente insufficiente per rafforzarne gli organici; sicuramente non mancano i progetti innovativi che, se realizzati e valorizzati adeguatamente, potrebbero davvero consentire uno sviluppo duraturo per il futuro del Paese. Tuttavia è opportuno che il *recovery plan* includa al suo interno ulteriori progetti fondamentali per il rilancio del Mezzogiorno, come il potenziamento strategico del porto di Gioia Tauro e la valorizzazione dei territori tramite un piano di assunzioni nella pubblica amministrazione rivolto principalmente ai piccoli Comuni del Mezzogiorno, che sono stati esclusi dal piano delle assunzioni. Pertanto, signora Ministra, in conclusione le chiedo di sapere quali altre iniziative intende promuovere per sanare il divario tra Nord e Sud e fare in modo che il Mezzogiorno possa trasformarsi nel volano di un nuovo sviluppo. se il ministro Brunetta, provvedendo a un aumento del numero e dei profili assunti, darà la possibilità di attivare convenzioni con ordini professionali e università per supportare gli enti locali del Sud e metterli al passo con il resto del Paese.

mancava un capitolo esplicito dedicato al Sud e si faceva del Mezzogiorno un obiettivo trasversale alla programmazione del PNRR. Affinché questa trasversalità non fosse elusiva del problema Mezzogiorno, nell'attuale nuova versione del PNRR ci sarà un vero e proprio capitolo Sud. Nella Conferenza unificata, cui a breve parteciperò, potrò dedicare più tempo all'illustrazione del valore della quota Sud compresa all'interno del Piano. Una novità qualificante che abbiamo introdotto nella nuova versione del piano è la riforma e i relativi investimenti delle zone economiche speciali. La misura prevede un pacchetto di interventi per 600 milioni di euro per le infrastrutture delle aree retroportuali e connesse, una robusta semplificazione amministrativa e un incentivo più intenso per gli investimenti nei beni strumentali. Questa linea di intervento non era ricompresa nella precedente stesura del piano. Tra i principali interventi su cui poi il Ministero per il Sud sta concentrando la sua attenzione ci sono i cosiddetti ecosistemi dell'innovazione. Agli 1,3 miliardi previsti su base nazionale dal Ministero dell'università e della ricerca, e dunque in parte da territorializzare al Sud, aggiungiamo, con la componente interventi speciali di coesione, ulteriori 350 milioni. L'obiettivo è quello di replicare su più aree del Mezzogiorno l'esempio virtuoso e positivo del polo di innovazione di San Giovanni a Teduccio, dove ricerca e imprese innovative stanno davvero cambiando le sorti di un territorio difficile. Questi e altri investimenti necessitano - è innegabile - di una pubblica amministrazione efficiente. A questo proposito sono consapevole che la procedura selettiva appena avviata con il ministro Brunetta per assumere 2.800 tecnici nel Mezzogiorno rappresenti soltanto un primo passo, per quanto significativo. Non vi sarà poi sfuggita l'adozione di una procedura lampo attraverso un concorso unico nazionale che ci consentirà di assumere, nel giro di cento giorni, questi 2.800 giovani professionisti che andranno a irrobustire la capacità progettuale delle amministrazioni del Sud, che da questo punto di vista sono più carenti e deficitarie rispetto alle amministrazioni del Centro-Nord. Naturalmente l'obiettivo immediatamente successivo, cui stiamo lavorando in sinergia con il ministro Brunetta, è quello di mettere in campo in tempi brevi ulteriori interventi su vari fronti, sia di carattere stabile che come supporto a specifiche azioni di sviluppo per il Sud.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

che finora ha penalizzato l'intera offerta imprenditoriale presente in questa parte d'Italia, costringendo anche le risorse migliori a fuggire dall'isolamento lavorativo, esautorando le potenzialità dei nostri territori che, senza gioventù e spunti e spunti di rinnovamento hanno perso negli anni anche la forza di autosostenersi, puntando sull'esistente. L'obiettivo unico che condividiamo con lei è restituire al Sud Italia quella coesione culturale ed economica che oggi può essere raggiunta con un utilizzo attento del *recovery plan*. Riteniamo che, in quest'ottica, la leale collaborazione politica sia l'unica chiave possibile per recuperare la credibilità che meritiamo, non solo in tutta Italia ma anche a livello mondiale.

il collega Dario Stefano e il sottoscritto, a nome del Gruppo PD, pongono con questa interrogazione il dito sulla piaga. Dico, senza retorica, che la presenza di asili nido nel Mezzogiorno è la piaga e, forse, l'elemento più significativo e drammatico della spaccatura dell'Italia. È l'elemento che frena la crescita del Mezzogiorno, che condiziona negativamente lo sviluppo cognitivo, relazionale, umano del bambino nel Mezzogiorno e frena la pari opportunità di genere, perché penalizza soprattutto le donne. Siamo ben lungi dal centrare gli obiettivi europei di Barcellona: garantire almeno al 33 per cento dei bambini sotto i tre anni un posto in asilo nido

Non c'è misura più efficace, per decriptare il grado di civiltà di un popolo, di una rete diffusa, adeguata e gratuita di nidi e servizi per l'infanzia. La pandemia ha aggravato pesantemente questa carenza. So bene che è nella sua sensibilità e in quella del Governo tale questione ed è per questo che le chiediamo, col collega Stefano e col Gruppo PD, una decisa e forte iniziativa politica, perché si utilizzi il fondo previsto dalla legge di bilancio 2020 e si preveda nel PNRR una specifica una specifica misura attuativa per potenziare la rete degli asili nido nel Mezzogiorno. Signor Presidente, onorevoli senatori, la legge di bilancio per il 2020 ha finanziato, tramite l'istituzione del Fondo asili nido e scuole dell'infanzia, progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido e scuole dell'infanzia, con priorità per strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane. Segnalo che, all'epoca, il Ministro per il Sud non venne incluso tra i Ministri concertanti per stabilire, tra l'altro, i criteri di riparto delle modalità di utilizzo di quelle risorse, nonostante, tra gli obiettivi principali della disposizione, vi fosse, non solo il miglioramento del quadro delle aree svantaggiate, ma anche la riduzione degli squilibri territoriali, che costituisce il compito primario del Ministero per il Sud. Per questa ragione, rassicuro gli onorevoli interroganti, rendendo noto che, pur non avendo potuto partecipare alle scelte sulla concreta ripartizione delle risorse previste da quel Fondo, ho chiesto e ottenuto puntuale rassicurazione dal Ministero dell'istruzione che, alle aree svantaggiate di cui il Sud rappresenta la maggioranza, è stata destinata una percentuale non inferiore al 60 del complesso degli interventi. Questa riserva non esclude che i Comuni del Mezzogiorno possano concorrere all'attribuzione delle risorse complessive anche del restante 40 per cento. In tal senso, ribadisco in questa sede la mia volontà, già manifestata ai Ministri concertanti, di intervenire quanto prima con una modifica normativa, che includa il Ministro per il Sud tra i componenti della cabina di regia istituita per il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti. In tal modo, nella fase di concreta esecuzione delle misure, potrò avere la consapevolezza di quanto davvero sarà destinato al Mezzogiorno. Accanto a questo, nei prossimi giorni, si terrà la prima seduta della cabina di regia del protocollo d'intesa tra il Ministero per il Sud e Cassa depositi e prestiti, tra i cui obiettivi abbiamo espressamente previsto il sostegno progettuale di Cassa depositi e prestiti all'edilizia scolastica di prima infanzia nei Comuni. Il tema dei nidi, senatore Pittella, come lei ha avuto modo di affermare nel corso del suo intervento, è di assoluta priorità e rappresenta il presupposto ineludibile per affrontare seriamente il dibattito sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, che considero come noto - cruciale per assicurare il vero rilancio del Mezzogiorno e delle aree svantaggiate, ma anche cruciale per superare quel divario di cittadinanza inaccettabile in un Paese civile come il nostro impedisce ai cittadini meridionali l'accesso ai diritti fondamentali, a cominciare da asili nido, istruzione, mobilità, trasporti e sanità. Su questo *dossier* il Ministero per il Sud è impegnato e conto di potervi dare notizie riguardo alle iniziative che assumeremo nelle prossime settimane. ringrazio, Ministra, anche a nome del collega Stefano. Churchill diceva che la parola è l'unica cosa che dura per sempre. Per noi la sua parola vale, anche se siamo di fronte ad una contraddizione tipica del nostro Paese del Ministero del Sud nella cabina di regia su questa materia. Noi pertanto appoggeremo la modifica di questa norma assurda. Colgo l'occasione, oltre che per ringraziarla per gli impegni presi, per dirle attenzione a come si muove il *recovery fund* sul Mezzogiorno e a garantire le gambe al Mezzogiorno, perché utilizzi i fondi previsti. Attenzione alla coda dei programmi dei fondi strutturali e alla nuova programmazione degli stessi, anche in rapporto ai servizi da dare alle donne e all'infanzia. Attenzione alla strategia nazionale sulle aree interne e alla situazione drammatica in cui vivono i Comuni che soffrono lo spopolamento. Le segnalo un disegno di legge del Gruppo PD, di cui sono primo firmatario, che aiuta a ripopolare questi Comuni. È una grande questione di democrazia.

Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, nell'ambito del Next generation EU, che l'Unione Europea ha offerto ai Paesi membri per uscire dall'emergenza economica, oltre all'ormai stranoto *recovery fund*, c'è anche il fondo React-EU; un fondo di cui si parla poco, ma che è molto importante, perché è corposo (per l'Italia vale circa 13 miliardi di euro) e perché è disponibile in tempi brevi. Parliamo di uno strumento che sicuramente potrà rappresentare un sostegno molto importante per il nostro Mezzogiorno, ancor più in questo momento storico, e per questo va programmato con grande attenzione, responsabilità e tempestività. Con il React-EU si potranno finanziare gli interventi più urgenti e sarà possibile assicurare il dovuto aiuto a tutte quelle imprese messe messe in ginocchio dalla pandemia. Di questi 13 miliardi di euro, infatti, sappiamo che circa 8,36 dovrebbero andare al Sud e sono destinati a misure molto importanti, come la fiscalità di vantaggio, i *bonus* per le assunzioni di giovani e donne, il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e la loro digitalizzazione, la transizione energetica e l'economia circolare. Le risorse andranno anche alla trasformazione digitale della didattica scolastica, alla riduzione delle tasse universitarie e al comparto della sanità. Di queste, fatto non trascurabile, ben 136 milioni dovrebbero essere destinati all'acquisto di vaccini. Nel complesso, quindi, il React-EU potrà essere una vera e propria boccata di ossigeno immediata per le Regioni meridionali, una leva fondamentale per la ripresa economica di quei territori. La fiscalità di vantaggio, per esempio, è una misura fondamentale per rilanciare il Sud ed è uno dei tasselli di un mosaico complessivo necessario a sostenere le imprese, assieme alla semplificazione burocratica e alla riduzione strutturale delle imposte. Importante in tal senso sarà anche trattare fin da subito con

anche una sua conferma ufficiale), quali siano gli interventi previsti e con quale criterio saranno distribuiti tra le diverse Regioni del Mezzogiorno. territoriale*. Ringrazio la senatrice Giammanco per aver portato all'attenzione di questa Assemblea la programmazione legata al React-EU. Il programma React-EU, previsto nell'ambito del Next generation EU, destina risorse aggiuntive per la politica di coesione 2014-2020 indirizzate ai Paesi più colpiti dalla pandemia. Dei 47,5 miliardi complessivi, il nostro Paese beneficia della quota più alta, 13,5 miliardi. Lo scorso 9 aprile ho provveduto a inviare alla Commissione europea il documento di programmazione del piano React-EU, con l'indicazione puntuale delle linee di intervento elaborate all'esito di un accurato percorso istruttorio. Abbiamo ottenuto la quota più alta dei fondi del React-EU, quindi avevamo il dovere di essere tra i primi in Europa e tra i più concreti nel definire la programmazione per spenderli e sono soddisfatta perché ci siamo riusciti. Il piano inviato alla Commissione, rispetto alle bozze precedenti, valorizza innovazione *green*, introduce un nuovo capitolo per affrontare il cronico problema degli acquedotti colabrodo, irrobustisce i sostegni alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e investe risorse nel campo della ricerca, dell'istruzione primaria e secondaria e del lavoro. Abbiamo puntato esclusivamente su misure effettivamente realizzabili entro la scadenza del 2023, gestite a livello nazionale attraverso lo strumento dei PON. Al Mezzogiorno sono destinati circa i due terzi dell'intero pacchetto, per un ammontare pari a quasi 8,5 miliardi. La decontribuzione dei contratti di lavoro al Sud assorbe da sola 4 miliardi, ma sono destinate alle Regioni meridionali altre importanti risorse: 313 milioni per interventi di riduzione della dispersione idrica delle reti; 750 milioni su 1,5 miliardi del Fondo nuove competenze e altre politiche attive del lavoro; 400 milioni su 500 del Fondo garanzia piccole e medie imprese; 100 milioni su 200 del Fondo green venture capital; 57 milioni per il potenziamento degli istituti agrari e ancora interventi per la connettività e la digitalizzazione delle aule scolastiche. Oltre 2 miliardi del Piano hanno come obiettivo trasversale la sostenibilità ambientale, tanto al Sud come al Centro-Nord. Direi che il React-EU rappresenta un banco di prova importante per il nostro Paese, è un po' la prova generale del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È il primo strumento su cui l'Italia può e deve dimostrare capacità di programmazione da un lato e certezza dei tempi di investimento dall'altro. Sulla capacità di programmazione, credo che abbiamo dato una prova di tempestività e speriamo anche di efficienza, sta ai vari livelli di Governo centrale, regionale e anche locale fare altrettanto nella realizzazione delle opere. *(FIBP-UDC)*. Ministro, la ringrazio per la risposta, di cui mi ritengo molto soddisfatta. Lei sa bene che le potenzialità del Sud sono incredibili, ma che serve superare la questione meridionale e quindi affrontarla, una buona volta, come questione nazionale. Viviamo in un Paese spaccato, bisogna agire in fretta e il React-EU ci dà la possibilità di dare risposte immediate ai cittadini meridionali. I ristori sono una misura sacrosanta e necessaria, ma pur sempre emergenziale. Compito del Governo deve essere colmare il divario economico, sociale e occupazionale tra Nord e Sud del Paese, un divario che - ahimè - con la pandemia pandemia è ulteriormente aumentato. Per questo mi auguro che l'opportunità offerta dal React-EU venga colta, così come quella rappresentata dal Fondo di sviluppo e coesione, Ministro, perché non è accettabile che nei sette anni di programmazione 2014-2020, dei 73 miliardi di dotazione complessiva del fondo sia stato speso solo poco più del cento. La invito anche a vigilare affinché, nella versione definitiva del PNRR, venga effettivamente rispettato il vincolo del 34 per cento per le risorse complessive del *recovery fund* da destinare al Sud *(Applausi)*, in modo da evitare che nei conteggi finali siano sovrapposte e computate anche risorse

vada assolutamente incrementata. Si ritiene infatti opportuno fissare una destinazione di risorse che sia almeno parzialmente coerente con i criteri di ripartizione delle risorse che l'Unione europea ha destinato agli Stati membri: Stati membri: popolazione, inverso del PIL *pro capite* e tasso di disoccupazione. Sempre nella relazione, si raccomanda poi la prioritaria definizione dei LEP, da lei appena citati, tra le riforme strutturali del PNRR. Ciò al fine di recuperare i divari nella fornitura di servizi pubblici essenziali, affinché si possano esercitare pienamente i diritti civili e sociali. Le stesse osservazioni sono state ribadite anche nella relazione della Camera dei deputati, con un'aggiunta: l'aggiustamento dei criteri di ripartizione non deve considerare le risorse per interventi in essere, cioè non deve considerare quelle risorse che sono già incluse nei tendenziali di finanza pubblica, cioè nel React-EU. Ministro, in occasione della sua audizione avvenuta in Senato il 16 marzo scorso presso le Commissioni 5a e 14a, posi alla sua attenzione proprio questi temi e le chiesi se il Governo avesse inteso adottare gli stessi criteri di riparto.

è stata posta anche da alcuni amministratori locali, come i Presidenti di Regione, in occasione degli importanti stati generali da lei indetti, e da ben 500 sindaci che aderiscono alla rete Recovery Sud. Tali amministratori locali hanno scritto al Presidente della Commissione europea europea chiedendo una maggiore tutela per il Sud e un'attenta vigilanza sull'utilizzo dei fondi. Il timore è infatti quello di andare incontro a un diretto intervento dell'Unione europea che, lo ripeto, ha disposto per l'Italia una quota importante di risorse, proprio in considerazione dei criteri appena elencati. Pertanto, le chiedo nuovamente se il Governo intenderà applicare il criterio di riparto richiesto nelle suddette relazioni parlamentari e, come chiesto nelle suddette relazioni, se il Governo intenderà definire i LEP. LEP. Chiedo a lei esplicitamente se ritenga corretto che i diritti costituzionali possano essere finanziati con risorse straordinarie europee e non con fondi nazionali ordinari (mi riferisco ai LEP). Infine, le chiedo qual è la quota esatta di risorse che complessivamente il Governo intende destinare al Mezzogiorno, al netto dei fondi estranei alle dotazioni del Next generation UE. Signor Presidente, onorevoli senatori, con riguardo alla quota Sud nel PNRR e alla necessità di superare, così come sollevato dall'onorevole interrogante, la percentuale del 34 per cento di investimenti nel Mezzogiorno - necessità rilevata anche nelle relazioni a cui la senatrice Ricciardi ha fatto riferimento posso rassicurare che questa è stata la priorità assoluta su cui, sin dai primi giorni del mio Ministero, ho concentrato la mia attenzione. D'accordo con il ministro Franco, abbiamo avviato un lavoro di ricognizione volto a costruire uno specifico capitolo Sud che non c'era, come ho ricordato nel corso della replica alla prima interrogazione - attraverso un lavoro non solo di difesa, ma anche di incremento degli interventi dedicati al Mezzogiorno. In virtù di questo lavoro e grazie al lavoro di difesa, ma soprattutto di incremento, la quota Sud oggi arriva al 40 per cento, una cifra - lo voglio sottolineare - a cui con ogni probabilità non saremmo arrivati senza un'attenta attività di verifica, misura per misura, svolta da tutti i Ministeri coinvolti, e di implementazione delle diverse missioni. Non lo dico per mettere le mani avanti, ma non vi sfuggirà che un conto è lavorare al più grande piano di ricostruzione per il nostro Paese dal dopoguerra in poi, avendo un orizzonte temporale di un anno, e un altro conto è riuscire a farlo avendo due mesi di tempo. Personalmente, nella mia visione avrei costruito un capitolo Sud, dedicato agli interventi al Sud, sin dall'inizio, sin dalla prima stesura del Piano, ma sono stata costretta a lavorare sull'impostazione che mi sono trovata. A breve, nel mio intervento in Conferenza unificata, avendo più tempo potrò entrare nel dettaglio delle singole missioni. Cito solo, a titolo di esempio, per la particolare rilevanza della missione, quella dedicata a "Infrastrutture per una mobilità sostenibile", caratterizzata dall'avere la quota Sud più rilevante, il 52 per cento. L'alta velocità ferroviaria nel Mezzogiorno è la vera protagonista di questa missione, con il finanziamento dei lotti funzionali, delle linee Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Messina-Catania, Roma-Pescara e Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia. può salire oltre il 40 per cento, se aiuteremo gli enti territoriali e le imprese a competere ad armi pari con quelle del resto del Paese, e cioè ad assorbire una quota maggiore delle risorse che saranno messe al bando. Ci sono alcune misure, come per esempio l'ecobonus, che storicamente non sono adeguatamente assorbibili dal Mezzogiorno, quindi stiamo lavorando a modifiche normative che possano rendere il Sud capace di attrarre queste importanti risorse. Quanto al tema dei LEP, che considero centrale per lo sviluppo del Mezzogiorno, per la riduzione degli squilibri territoriali tra Nord e Sud e per garantire l'accesso di tutti i cittadini ai servizi fondamentali indipendentemente dal luogo di residenza, sono al lavoro con i Ministri competenti per accompagnare l'adozione del PNRR con una puntuale definizione con norma primaria dei livelli essenziali delle prestazioni. Partiremo dalla prima infanzia, cioè dagli asili nido, e dal sociale, con un'impostazione che tenga conto dei diversi livelli di partenza nelle realtà del Paese e dei contenuti qualitativi, e non solo quantitativi, delle prestazioni che si forniscono e della necessità di sostenere queste azioni con risorse nazionali che ogni anno siano appositamente destinate con legge di bilancio.

assolutamente ripartire dal PNRR e, in assenza di una vera coesione sociale e territoriale, tutto ciò non si può avere, se non definendo i LEP e rifinanziando grandi opere, così come ha promesso in questo momento. Tengo anche a sottolineare che la Svimez ha stimato che investire nel Mezzogiorno il 50 per cento dei fondi Next generation EU comporterebbe un incremento del PIL meridionale dell'11,6 per cento e questo non lo dico io, ma istituti di ricerca e la stessa Banca d'Italia confermano che investire nel riequilibrio territoriale alimenterebbe un effetto indiretto sulla produzione del Centro-Nord. Per esempio, un euro investito al Sud genera 1,3 euro di valore aggiunto per l'intero Paese, grazie ad un effetto moltiplicatore degli investimenti pubblici in queste aree. Un'ultima cosa: il Covid ha messo a nudo uno spaccato del nostro Paese; dal 2002 al 2017, due milioni di cittadini hanno abbandonato il Sud, per lo più giovani, il 33 per cento dei quali laureati. In quindici anni, il Mezzogiorno ha perso lo stesso numero di residenti della città di Roma. Dico questo nella consapevolezza che, se riparte il Meridione, riparte l'Italia.

signora Ministra, purtroppo l'Italia sta tornando a essere di nuovo meta privilegiata per la migrazione di migliaia e migliaia di disperati, soprattutto migranti economici, che arrivano costantemente sulle nostre coste. Come è a lei ben noto, nei primi mesi di quest'anno gli sbarchi sono più che raddoppiati rispetto al 2020, nello stesso periodo, e più che duplicati rispetto allo stesso periodo del 2019: una vera e propria invasione, che crea enormi problemi, soprattutto in un momento grave di emergenza come quello rappresentato dalla pandemia, aggravato dal fatto che molti di questi immigrati sembra strano - sono liberi di circolare liberamente sul territorio nazionale, a differenza di tutti gli italiani e di tutti gli immigrati regolari, con il rischio di diffondere il contagio e, in particolare, di portare in Italia varianti del virus resistenti anche alle cure e ai vaccini. È altrettanto noto che infiltrati in questa massa di disperati ci sono anche molti affiliati alle varie mafie straniere, che stanno prendendo il controllo di gran parte delle nostre periferie, e purtroppo, in alcuni casi, è stata riscontrata anche la presenza di terroristi. Come ben sa, grazie al lavoro coraggioso di alcune procure e di alcuni magistrati, si è scoperto ciò che in realtà già si sapeva, e cioè che le ONG, lungi dallo svolgere semplicemente un lavoro di recupero dei dei naufraghi nel Mediterraneo, molto spesso svolgono un ruolo di sostegno e ausilio ai trafficanti di carne umana e di esseri umani. In alcuni casi, sono addirittura complici di questo traffico indegno.

priva di regole e di controllo, che rischia di creare all'Italia e gli italiani ancora più sofferenze di quelle che già purtroppo stanno patendo in questo periodo. Signor Presidente, onorevoli senatori, i flussi migratori provenienti dal Nord Africa sicuramente rappresentano importante, che seguiamo con la massima attenzione. Ritengo che innanzitutto sia necessaria la disarticolazione dei sodalizi criminali che certamente portano alla perdita di vite umane. È quindi sicuramente necessario contenere - ne siamo certi e stiamo facendo tutto il possibile - l'immigrazione illegale. Un efficace contrasto del traffico dei migranti e della tratta richiede due condizioni: in primo luogo, serve un approccio condiviso con i Paesi terzi di origine sul transito dei flussi, che devono cooperare ed essere sostenuti nella costruzione di efficaci sistemi di controllo delle frontiere; in secondo luogo, occorre il rilancio della dimensione esterna della politica migratoria europea, come ho avuto modo di rimarcare in occasione della riunione congiunta dei Ministri degli esteri e dell'interno svoltasi il 15 marzo scorso. Occorre, in definitiva, anche uno sforzo straordinario dell'Unione europea per rilanciare il dialogo politico e gli accordi di partenariato con i Paesi terzi, in modo da prevenire i flussi migratori, facilitare le attività di rimpatrio e, nel contempo, intensificare la cooperazione nel campo dello sviluppo economico sostenibile e della migrazione legale. Tale versante delle politiche migratorie richiede un maggior coordinamento tra gli organismi di Governo dell'Unione europea e i Paesi membri e, in tale contesto, l'Italia è pronta a offrire un contributo concreto. Passando alla dimensione operativa, uno strumento importante di controllo delle frontiere marittime esterne è costituito dall'operazione di pattugliamento congiunto Themis, condotta sotto l'egida di Frontex, tuttora in corso, finalizzata alla sorveglianza marittima per il controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale. Inoltre, attraverso l'impiego dei finanziamenti europei previsti dal Fondo di sicurezza 2014-2020, è stato realizzato l'ammodernamento della rete *radar* costiera della Marina militare e della della Guardia di finanza, proprio per potenziare la capacità di intercettamento in mare anche di imbarcazioni piccole utilizzate dai migranti per raggiungere le coste italiane. Circa i rischi sanitari connessi ai flussi migratori evocati dall'onorevole interrogante, vorrei precisare che tutti i migranti giunti sul territorio nazionale, prima del loro inserimento nel circuito dell'accoglienza, sono sottoposti ai protocolli sanitari finalizzati al contenimento del contagio del contagio da Covid e regolarmente svolgono un periodo di quarantena. Scendono dalle navi, dove svolgono il periodo di quarantena, soltanto dopo aver fatto il tampone con esito negativo. Quanto all'attività di prevenzione del rischio di infiltrazione terroristica nei flussi migratori, le forze di Polizia mantengono un elevato livello di attenzione. In quest'ambito operano apposite *task force* composte da esperti antiterrorismo dell'immigrazione, attive nelle principali aree di sbarco e negli *hotspot* nazionali, con il compito di analizzare proprio la possibilità di infiltrazioni terroristiche. Signora Presidente, signora Ministra, purtroppo non posso dichiararmi soddisfatto della sua risposta, perché queste attività che ha elencato in modo dettagliato (cosa di cui la ringrazio) erano in essere anche uno, due o tre anni fa. Cos'è cambiato rispetto ad allora? Perché i flussi migratori sono decuplicati in questo periodo? La risposta è semplice: perché a dicembre scorso sono stati smantellati i decreti sicurezza. Lei lo sa bene, in quanto era la prima firmataria di quel disegno di legge. Avete trasformato in modo colpevole l'Italia in una meta privilegiata per gli immigrati; avete attaccato attaccato un manifesto, in tutto il Terzo mondo, in base al quale qui si può arrivare e si è accolti. Bisognerebbe fare come in Spagna. Cos'ha fatto la Spagna? la Spagna? Ha fatto una regola molto semplice, che è stata riconosciuta legittima dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con una sentenza dello scorso anno: anno: ha fatto in modo che chi davvero ha diritto all'asilo possa fare domanda presso le ambasciate del Paese di origine o anche del Paese di transito. Chi vuole venire fa domanda in ambasciata o in consolato e, se ha diritto, viene; tutti gli altri vengono respinti. La Spagna, che pure è un paese dell'Unione europea, respinge in massa i migranti, perché consente loro di venire regolarmente, senza correre il rischio di rimetterci la vita e di essere sfruttati

sì che non sia sfruttata in modo indegno è quello di impedire le partenze. Questa è l'unica strada che, secondo noi e secondo Fratelli d'Italia, è percorribile. *(Applausi)*.

1976, n. 752, ha introdotto gli esami di bilinguismo per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca finalizzato al rilascio, da parte delle commissioni, di 4 tipi di attestato a seconda del livello di conoscenza delle lingue italiana e tedesca (C1, e tedesca (C1, B2, B1 e A2); l'indennità di bilinguismo è calcolata con riferimento all'attestato richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione stessa; Considerato che l'articolo 1 del decreto legislativo n. 95 del 2017 ha sostituito l'articolo 6 del decreto del innalzando il livello rispetto al titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli di base della Polizia di Stato, da diploma di istruzione secondaria di primo grado a diploma d'istruzione secondaria di secondo grado; a seguito dell'innalzamento del requisito rispetto al titolo di studio richiesto, i soggetti interessati hanno inoltrato domanda alla Questura di Bolzano di allineamento dell'indennità di bilinguismo in busta paga, come previsto dalla normativa in vigore, dal livello "B1" al livello "B2", con richiesta di corresponsione dei relativi arretrati economici maturati; tali domande risultano, allo stato attuale, inevase presso gli uffici competenti, si chiede di sapere quali siano le ragioni del ritardo nella presa in carico delle domande di allineamento dell'indennità di bilinguismo secondo i nuovi livelli stabiliti e se il Ministro in indirizzo non intenda sollecitare gli uffici competenti al disbrigo di tali domande.

occorre premettere al riguardo che la corrispondenza tra il livello di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca e il titolo di studio richiesto per l'esercizio della funzione amministrativa

Questa normativa prevede che l'indennità di seconda lingua sia calcolata con riferimento ai vari gradi degli attestati di conoscenza linguistica e non rapportata alla funzione ricoperta e che, qualora il livello di conoscenza linguistica conseguito sia più elevato rispetto al grado richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale ricoperta, l'indennità debba essere calcolata con riferimento al livello richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale.

è stato innalzato il titolo di studio per l'assunzione degli agenti della Polizia di Stato dal diploma di istruzione secondaria di primo grado al diploma di istruzione di secondo grado. Tuttavia, in ossequio al principio *tempus regit actum*, deve trovare applicazione ai dipendenti la normativa vigente alla data del loro ingresso nella Polizia di Stato, non potendo giovarsi coloro che sono entrati successivamente della modifica intervenuta Questo orientamento, peraltro, è stato anche condiviso dalla più recente giurisprudenza amministrativa, tant'è che il TAR sezione di autonoma di Bolzano, la sentenza n. 269 del 6 novembre 2019, ha statuito che la circostanza che il ricorrente sia in possesso di un attestato di bilinguismo di grado più elevato rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione non determina il diritto a percepire l'indennità corrispondente, ostandovi il chiaro disposto del quinto comma dell'articolo 1 del citato comunque assicurare che la questione è all'attenzione dei miei uffici e verranno fatti tutti gli approfondimenti necessari, all'esito dei quali saranno adottati i provvedimenti conseguenti.

proprio per facilitare l'uso della lingua tedesca nei rapporti fra il cittadino e le Forze dell'ordine, soprattutto nel nostro territorio.

intraprendere per contrastare il rischio concreto di infiltrazioni della malavita nel tessuto economico, sociale e politico del territorio napoletano, già investito da un pesante disagio, anche a seguito dell'emergenza sanitaria ed economica. L'attenzione di questo mio intervento odierno riguarda due città dell'area napoletana: Castellammare di Stabia, che ha più di 60.000 abitanti, dove il *clan* D'Alessandro è presente da tre generazioni, e Torre del Greco, che ne ha 85.000. In entrambi i Comuni inchieste della magistratura e indagini delle Forze dell'ordine evidenziano l'interesse dei *clan* non solo nel sistema degli appalti pubblici, ma anche nella politica locale. Le ricordo che a Castellammare di Stabia a marzo sono stati arrestati 16 esponenti del *clan.* La cosca avrebbe messo le mani nella sanità stabiese. Sa anche che sono state riaperte le indagini su due omicidi eccellenti di Castellammare: quello di Sebastiano Corrado, consigliere comunale dell'allora Partito Democratico della Sinistra, e quello di Luigi Tommasino, eletto in Comune proprio nel Partito Democratico. Le sono chiari quindi l'intreccio tra la politica locale e la camorra e, di conseguenza, la necessità di combattere le opacità. C'è poi Torre del Greco: anche qui, il quadro che emergerebbe da un'indagine che già nell'aprile 2019 aveva condotto all'arresto di diversi soggetti, se confermato, lascerebbe trasparire una regia unica e ben definita volta a condizionare in maniera inequivocabile e criminale il voto delle elezioni amministrative del 2018 su più fronti. Insomma, signora Ministro, non ritiene il caso di istituire le commissioni d'accesso nei due Comuni per verificare le eventuali infiltrazioni dei *clan* della camorra? si fa riferimento al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nei Comuni di Torre del Greco e Castellammare di Stabia. L'onorevole interrogante chiede di sapere se in relazione a tali amministrazioni si intenda o meno attivare il potere di accesso di cui all'articolo 143 del testo Con riferimento al Comune di Castellammare di Stabia, lo scorso 25 marzo è stata depositata un'ordinanza cautelare in carcere nei confronti di 16 esponenti di spicco del *clan* D'Alessandro, in cui sono state ipotizzate ingerenze della criminalità organizzata in appalti pubblici riferiti anche all'ospedale San Leonardo. Tale quadro investigativo è stato oggetto di esame da parte del prefetto di Napoli, che, dopo una prima immediata riunione di coordinamento interforze, ha approfondito la questione in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi il 9 aprile scorso, a cui ha partecipato anche il procuratore distrettuale della Repubblica. In tale occasione si è convenuto che il contesto di Castellammare di Stabia vada monitorato con la massima attenzione, anche attraverso l'attivazione di straordinari servizi di controllo del territorio e che il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata venga ulteriormente approfondito da parte delle Forze di polizia per verificare la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo 143 del TUEL. Il prefetto di Napoli a tal riguardo mi consegnerà a breve una relazione, in esito alla quale poi si valuterà il caso e se fare o meno l'accesso presso quel Comune, esercitando quindi i poteri di accesso. Per quanto riguarda lo scenario criminale di Torre del Greco, la notte del 1° aprile, come evidenziato nell'interrogazione, è stata data esecuzione, anche qui da parte dell'Arma dei carabinieri, alla misura cautelare personale emessa il 26 marzo scorso dal gip di Torre Annunziata, sottoponendo agli arresti domiciliari, tra gli altri, un consigliere del Comune. Tali misure sono state disposte nell'ambito di una più ampia e articolata indagine, con la quale si è accertato che in occasione della consultazione amministrativa del 2018 tutti gli indagati avrebbero fatto parte di un'associazione criminale finalizzata alla compravendita di voti. Anche la situazione del Comune di Torre del Greco è stata oggetto di approfondimento nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla prefettura di Napoli del 9 aprile e, in quella circostanza, nel prendere atto della richiesta avanzata dallo stesso sindaco del comune di Torre del Greco di inviare la richiesta per una commissione d'accesso presso il proprio Comune, si è convenuto sull'esigenza che gli elementi informativi siano oggetto di approfondimento da parte delle Forze di polizia, fine di valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per attivare le procedure stabilite dall'articolo Anche per tale amministrazione comunale sono pertanto in attesa degli elementi che mi fornirà il prefetto di Napoli all'esito del comitato, per poi decidere se esercitare i poteri di accesso.

sa, proprio pochi giorni fa una delegazione di parlamentari napoletani del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle, insieme al sottoscritto, ha incontrato il dottor Marco Valentini, il prefetto di Napoli. Tutti abbiamo colto l'impegno da parte della prefettura, del suo Ministero, delle Forze dell'ordine e della magistratura a fronteggiare l'emergenza criminale, sapendo che i fondi europei del *recovery fund* faranno gola alla criminalità organizzata. Non abbiamo altra strada che investire nella legalità per contrastare l'*escalation* della camorra, che si riproduce (nel caso di Castellammare di Stabia siamo infatti alla terza generazione di un *clan*), perché si relaziona con i poteri: con il potere politico, con quello economico e con quello finanziario. Per vincere bisogna recidere questi legami e soprattutto battere l'indifferenza. Premesso che: i flussi migratori provenienti dalla Libia nelle ultime settimane sono notevolmente aumentati:

che richiede misure supplementari di controllo e di isolamento che rischiano veramente di mandare il nostro sistema sapere quali azioni di politica interna ed estera, anche in accordo col Governo libico e con altri Paesi, stia programmando per impedire il continuo e incessante sbarco di migranti sulle nostre sulle nostre coste e, dall'altra parte, per collocarli equamente, magari dividendoli in tutta Europa, evitando che il nostro Paese, già pesantemente provato dall'emergenza sanitaria, sia ulteriormente gravato nell'affrontare problemi di ordine pubblico legati alla gestione dell'immigrazione clandestina.

respiro e collocate nel solco dei principi costituzionali e degli obblighi internazionali dell'Italia. A livello internazionale, in questi mesi l'aspetto principale delle politiche in materia di immigrazione il negoziato in corso a livello europeo per l'approvazione del Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Rispetto alle proposte contenute ho già avuto modo di chiarire nelle varie sedi anche europee la posizione dell'Italia. La nostra strategia negoziale si fonda sulla necessità del riconoscimento della specificità della gestione delle frontiere marittime, con sistemi di ricollocazione più stringenti per i migranti salvati in mare nel corso delle operazioni di ricerca e di soccorso, così come prevede l'accordo di Malta del 2019. Su tale strategia mi sono confrontata positivamente da poco, a Parigi, con il ministro Darmanin e presto lo faremo, congiuntamente al Ministro francese, con il ministro tedesco Seehofer. Sottolineo anche che stiamo facendo il massimo sforzo per far ripartire il meccanismo dei ricollocamenti, che è stato purtroppo bloccato dalla pandemia. L'altro punto cardine è l'affermazione di un equilibrio fondamentale tra responsabilità nella gestione delle frontiere esterne dell'Unione e solidarietà tra i suoi Paesi membri. Questa priorità è stata al centro dell'incontro ad Atene, lo scorso 20 marzo, in occasione del Med-5, un *Forum* informale che comprende comprende Italia, Grecia, Spagna, Cipro e Malta, cioè i cinque Paesi membri dell'Unione europea affacciati sul Mediterraneo e quindi fortemente esposti ai flussi come Paesi di primo ingresso. In questo quadro, ritengo essenziale collaborare con i Paesi di origine e transito dei flussi. In questo, l'Italia è impegnata nel processo di stabilizzazione, anche in Libia, delle istituzioni, in coerenza con il rapporto storico bilaterale che unisce i due Paesi. Uno sviluppo politico importante è la recente costituzione del Governo di unità nazionale, che dovrebbe condurre la Libia alle elezioni a dicembre. Conto di incontrare davvero a breve il mio omologo libico per ribadire la disponibilità italiana a un sostegno efficace e costruttivo.

sul fatto che bisogna essere operativi proprio con la Libia. Va bene tutta la normativa, ma occorre anche un accordo per cercare, appunto, sia di trovare una soluzione con

colleghi senatori, la situazione pandemica in Calabria, soprattutto nella provincia di Cosenza, peggiora di giorno in giorno, con un crescente aumento di contagi e di decessi: difficoltà nel contenimento e tracciamento del virus; strutture sanitarie ormai sature e al collasso; ricoveri bloccati; pazienti in fila al pronto soccorso; ambulanze in coda per ore davanti all'ospedale Annunziata di Cosenza; malati che purtroppo vi muoiono dentro, in attesa di essere ricoverati; personale stremato, chiamato a turni di lavoro massacranti; campagna vaccinale confusa e approssimativa, che procede a rilento, obbligando anziani e fragili, affetti da gravi patologie, ad affrontare per la prima dose di vaccino veri e propri viaggi della speranza a centinaia di chilometri di distanza. Le ataviche criticità della sanità calabrese, unite alla fallimentare gestione commissariale, che va chiusa definitivamente, rendono l'attuale situazione epidemiologica ancora più preoccupante in questa Regione da sempre in emergenza e che, com'era prevedibile, subisce l'urto della nuova ondata del virus, impreparata È giunto il tempo di archiviare questa deleteria pagina di espropriazione di diritti, autonomia e potere e di dare risposte ai calabresi. La sanità torni ai calabresi, stralciando il debito in capo allo Stato avviando subito una riorganizzazione complessiva della rete ospedaliera, con la riapertura dei presidi chiusi, con l'assunzione di più personale e con tutti i provvedimenti finalizzati a fermare l'emigrazione sanitaria. I sindaci, che, accogliendo l'appello del sindaco di Cosenza, il 17 aprile si ritroveranno davanti al pronto soccorso dell'ospedale civile di Cosenza, restano gli unici e soli avamposti dello Stato, a maggior ragione in una Regione già in ginocchio economicamente e socialmente, in affanno di suo nell'ordinarietà, figuriamoci nella straordinarietà di una pandemia dalle proporzioni di quella che stiamo vivendo. Sono vicino ai comitati civici, che hanno messo in campo un'azione di lotta che va sostenuta pacificamente. Vogliamo capire cos'è accaduto, cosa sta accadendo adesso in questa Regione e di chi sono le responsabilità. Mi aspetto dal Governo che finalmente anche alle cittadine e ai cittadini della Calabria sia garantita la piena realizzazione di un diritto primario sancito dalla nostra Costituzione: il diritto alla salute.

Uno dei mercati economici più fermi è da tempo quello dell'edilizia, un settore che più di ogni altro è trainante e moltiplicatore per una serie infinita di attori economici: penso ai progettisti, ai produttori di materiale edile, edile, elettronico e idraulico; penso ai muratori, agli intonachisti, agli imbianchini, ai rivenditori di materiali e così via, fino addirittura alle società immobiliari. È una catena lunga di cointeressati a questa economia e sta qui l'intelligenza legislativa ed economica del superbonus al 110 per cento, voluto e ideato dal MoVimento 5 Stelle durante il Governo Conte smuovere dalle fondamenta l'economia racchiusa attorno al più importante progetto che fa una famiglia normale, ossia costruirsi o comprare una casa. casa. Fatta questa premessa, vorrei denunciare qui in Aula un'anomalia, se non un'ingiustizia: il superbonus al 110 per cento sull'adeguamento sismico e l'efficienza energetica esclude le aree di ricostruzione del sisma del 1980 in Basilicata e Campania, o quantomeno è quello che appare da una presa di posizione della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate della Basilicata, la quale è dell'avviso che gli sgravi fiscali previsti dal decreto rilancio non sarebbero cumulabili con le agevolazioni già spettanti per le medesime finalità, sulla base di norme speciali, per interventi in aree colpite da eventi sismici. Cito l'organo di Confindustria, «Il Sole 24 Ore», del 2 marzo 2021: questi cittadini agevolati sulla ricostruzione del dopo-sisma del 1980 sarebbero esclusi anche dal miglioramento energetico delle loro abitazioni, su interventi delineati più di quarant'anni fa e senza tenere conto delle evoluzioni delle tecniche di interventi? La questione, signor Presidente, non è di poco conto, dato che il sisma del 1980 ha devastato due Regioni. In sostanza, si sta introducendo una rilevante disparità di trattamento tra i territori del Centro-Nord (Emilia Romagna, Abruzzo e Lazio), interessati da un sisma, e quelli del Sud Italia (Basilicata e Campania), colpiti dalla medesima tragedia. Credo che ci troviamo ampiamente dinanzi a una lacuna normativa, proprio per l'assenza di specifiche direttive riguardanti l'evento sismico del 1980, e abbiamo l'obbligo etico e sociale di porvi rimedio, per evitare che la tragedia della lunghissima e dolorosa ricostruzione delle aree del sisma del 1980 sia esclusa dalle agevolazioni della legge fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle. Serve un atto legislativo di interpretazione autentica del Ministero per chiarire che il divieto opera solo per eventuali pratiche di finanziamento in corso. Per questi motivi, ho depositato un'interrogazione e firmato l'emendamento del collega Santillo al decreto sostegni per porre riparo a tale grave *vulnus*, per il quale ci auguriamo giusta approvazione.

sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.